è intervenuto su questo provvedimento, al quale il Senato aveva apportato parecchie modifiche in termini sia di introduzione di nuovi articoli e nuovi commi che di stralcio o soppressione

Nonostante ciò, in questa seconda lettura alla Camera - la terza lettura in totale - ci sono state poche modifiche, molto circoscritte,

Senato. Parlerò di queste poche modifiche, dunque, perché il resto del testo non è oggetto della nostra trattazione, se non in sede di approvazione

adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore siano innanzitutto individuate e poi restino in vigore, benché risalgano al periodo rispetto al quale è stata prevista la loro abrogazione. È certamente un'esigenza Grazie si è ritenuto ovviamente che questo genere di leggi dovesse essere salvaguardato, come viene riportato anche nell'ultimo comma dello stesso articolo 4,

dove si specifica che i decreti legislativi in materia ambientale devono individuare le «caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e delle rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale

«un confronto con le regioni e gli enti locali che fossero interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali

la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e della Repubblica italiana; è un aspetto che in Senato avevamo considerato ovvio, ma che la Camera ha ritenuto di dover precisare. Ulteriori clausole sulla copertura sono contenute all'articolo 33, mentre all'articolo 34 viene estesa alle pubbliche amministrazioni regionali la facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata, in modo da sveltire le comunicazioni riguardanti le proprie attività d'ufficio. Altre misure in questo senso sono state introdotte all'articolo 35. Non ci sono altre modificazioni di rilievo,

Grazie

approfondimento sull'idoneità di questo intervento), nell'ambito del riassetto della disciplina del processo amministrativo, una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di poter avere una rapida risposta, compatibile con i tempi previsti dal procedimento elettorale, quando vi sia un contenzioso su questo

indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004», abolendo dunque casi particolari che erano stati introdotti.

al disegno di legge n. 1082-B per la parte che riguarda il codice di procedura civile sono abbastanza contenute nel loro numero e nel rilievo che hanno sul processo civile. In particolare, si è deciso che le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali non debbano essere decise con le norme fissate per le controversie in materia Uno dei punti che era stato a lungo discusso qui in Senato nella precedente lettura riguardava le testimonianze scritte.

al fallimento, in caso di presentazione di più proposte di di concordato, c'è stata una modifica che rende più agevole la soluzione dei problemi che si pongono. L'intervento della Camera è stato invece maggiormente significativo

Il primo comma del nuovo articolo 360*-bis* prevede che il ricorso sia inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. Il riferirsi ad elementi che possono confermare o mutare l'orientamento della Corte può apparire in qualche misura contraddittorio, perché perché *tertium non datur* (o conferma o muta), però il senso di questa norma, nella versione approvata in seconda lettura dal Senato, era formulata in chiave di ammissibilità, mentre ora, come ho detto, ci si riferisce invece alle ipotesi di inammissibilità. Questo potrebbe apparire ambiguo, ma l'ambiguità è agevolmente dissipata se si fa una più attenta lettura che conferisca un senso logico alla norma medesima, quindi una lettura necessitata e costituzionalmente corretta della previsione. In particolare, il ricorso sarà dichiarato inammissibile quando la decisione impugnata sia conforme alla giurisprudenza della Corte, a meno che - recita la norma - il ricorso non offra elementi per confermare o mutare l'orientamento della Corte stessa. Ora, mentre sul mutare significato è assolutamente chiaro, il riferimento al confermarlo potrebbe a prima vista sembrare illogico, posto che è ovvio che l'orientamento, se non si muta, non resta che confermarlo. quel decisivo riferimento resterebbe fuori della previsione in modo incostituzionale, data la funzione della Corte di cassazione; resterebbe fuori dunque un'ipotesi essenziale, quella secondo cui la Corte ritiene sì di confermare l'orientamento, ma con diverse motivazioni o anche solo con ulteriori e più ricche motivazioni, complementari ed esplicative di quelle precedentemente esposte, come tipicamente avviene quando la Suprema corte intende rispondere alle obiezioni provenienti dalla dottrina o comunque dai ricorsi che le vengono proposti. Con queste migliori precisazioni può meglio guidare la decisione dei giudici di merito. È evidente che il confermare deve intendersi seguito implicitamente dal riferimento a diverse o ulteriori motivazioni con cui supportare lo stesso *decisum* e quindi la stessa conclusione cui la Corte ha deciso sia giusto pervenire. Dunque, il ricorso non sarà ammissibile sempre, ma solo logicamente per mutare orientamento o per confermarlo, ma con differenti o ulteriori motivazioni.

in varie materie, per niente omogenee tra di loro. Si è detto da parte del Governo e della maggioranza che tali materie erano nei fatti tutte collegate dalla finalità di favorire lo sviluppo economico,

con il rischio di aver prodotto una legge onnicomprensiva che non ha consentito e non consente una riflessione seria approfondita su tantissimi argomenti, sui quali pure abbiamo cercato di dare, nelle varie Commissioni,

che hanno ampliato la sfera di intervento ancor di più e si è fatto ampio, troppo ampio, ricorso alle attribuzioni di delega. Tutto questo, nel suo insieme, sembra contraddire e suona in stridente contrasto con quanto previsto dal Capo II di questo stesso provvedimento ("Semplificazioni") e dall'articolo 3 ("Chiarezza dei testi normativi"). Tutt'altro, cari colleghi, si è prodotto in questo provvedimento. Alcuni riferimenti, per entrare nel merito. Si è modificata la legge Baccini del 2005, eliminandone alcune parti e abrogandone altre, talvolta in modo incomprensibile per gli stessi addetti ai lavori. Difficile rintracciare quale normativa preesista e quale rimanga in vigore. Difficile comprendere (parliamoci chiaro), anche da parte dei destinatari, in che cosa, quanto e come sia stata modificata la legislazione. la legislazione. Si mantengono parti della legge precedente. Per altre vi sono dei rimandi e dei richiami. Ci si troverà di fronte ad un ginepraio. Servirà l'ausilio di interpreti per uno studio approfondito. Si è intervenuti sulla legge n. 241 del 1990, modificandone pezzi, senza una visione di insieme,

almeno su di essa non si sia utilizzato il lavoro già svolto nella precedente legislatura, che aveva visto il concorso anche delle opposizioni e che poteva essere proficuo per chiarire meglio il testo normativo. Dunque, dove si poteva operare in modo articolato e più complesso si è scelto di procedere a pezzi. Si sono introdotte numerose deleghe, come ho già detto, le più rilevanti delle quali riguardano la semplificazione dei riti del processo civile, la conciliazione in materia civile e commerciale, la riforma del processo amministrativo, misure per lo sviluppo della banda larga. Relativamente alle singole disposizioni, si annoverano materie disparatissime: semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche;

Dal punto di vista del procedimento amministrativo, benché esso abbia effetto anche su chi fa parte della conferenza di servizi, si è disciplinato che taluni soggetti partecipino senza diritto di voto. Si è inoltre intervenuti sulla tutela del cittadino nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza delle Regioni e degli enti locali. Si sono introdotte deleghe al Governo (e qui la nostra battaglia esplicita alla Camera e al Senato è stata molto forte)

Si sono introdotte norme che riguardano le farmacie pubbliche e private per realizzare servizi socio-sanitari. Abbiamo insistito su questo per far comprendere come sia fondamentale - e con i nostri emendamenti abbiamo ottenuto qualche risultato risultato - rispettare le competenze delle regioni e i piani regionali. Si sono, inoltre, differiti i termini per leggi correttive ed integrative in materia ambientale; si è intervenuto sulla cooperazione internazionale, sui fondi FAS, sulla Corte dei conti, sugli enti locali, sulla pubblica amministrazione, sull'ENIT,

Non mi sembra un bel modo per affrontare le riforme di comparto! Queste norme, quindi, illeggibili e spezzettate ci impediscono di cogliere un'idea complessiva delle riforme in qualsiasi settore. Nel merito di tali norme abbiamo cercato con gli emendamenti di migliorare il testo, ma molte proposte ragionevoli ed articolate non sono state prese in considerazione.

Aumenteranno le complicazioni e noi siamo convinti che il lavoro in Commissione avrebbe prodotto un testo migliore ed anche in minor tempo. non avremmo sicuramente fatto mancare - come è dimostrato anche dalla presentazione di alcune nostre proposte - un apporto di merito costruttivo. Vorrei soffermarmi ancora sul tema delle deleghe, sollevato anche in corso d'opera nei nostri interventi. Nei fatti si è compiuto un travisamento del testo originale in una materia delicata come quella dell'attribuzione delle deleghe. Sappiamo da molte sentenze della Corte costituzionale ed anche dalla profonda ispirazione della nostra Costituzione che l'attività legislativa è fondamentalmente affidata al Parlamento;

finanziaria e che ha permesso di introdurre via via modifiche ordinamentali attraverso emendamenti, restringendo i tempi con determinate procedure su materie delicate, quale l'ambiente, la Corte dei conti (peraltro, di legge n. 847), l'Avvocatura dello Stato, la Carta nazionale dei servizi, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, il risparmio energetico e le norme sulla bancarotta.

sottraendo all'esame del Parlamento in modo puntuale intere parti che sono vere e proprie riforme ordinamentali e che qui sono passate come emendamenti. Ci chiediamo quale qualità della legislazione stiamo producendo;

comprensibili sia per il Parlamento che per i cittadini, affinché questi possano giudicare nel merito l'una o l'altra posizione su questioni rilevanti della vita del Paese e del territorio. Ecco, non viene fatto niente In contrasto con tante osservazioni prodotte da anni dal Comitato per la legislazione, ci troviamo di fronte ad un provvedimento costituito da un insieme di leggi, di richiami e di modifiche poco trasparente, in base alla semplificazione normativa, alla delegificazione, al cosiddetto Quando il Governo e la maggioranza vorranno confrontarsi seriamente su riforme organiche, troveranno - e hanno trovato, come è dimostrato - il contributo del Partito Democratico; tuttavia, quando si usa il potere del Governo e dei Regolamenti per umiliare il confronto nel Parlamento, per non favorire l'elaborazione di leggi chiare, noi non saremo mai d'accordo. Denunceremo, come abbiamo già fatto - ripeto - questo stato di cose che non è altro che lo specchio di un'insofferenza per la divisione dei poteri, principio cardine nelle democrazie moderne. Non è che non vediamo come la velocità delle decisioni, le pressioni sugli Esecutivi siano sempre più incalzanti. E, certo, sappiamo che questo tema è diverso rispetto a 20 o 30 anni fa. Ma questo significa allora affrontare seriamente il tema dei Regolamenti parlamentari, la riforma costituzionale. Già il tema dei Regolamenti potrebbe da solo produrre più celerità e non per questo meno elaborazione e contributo parlamentare. Ciò è stato dimostrato quando la volontà politica ha portato ad un confronto vero e costruttivo. trasformare il modo di lavorare delle Commissioni assegnando più importanza a questi luoghi nei quali il lavoro e il confronto di merito è molto più netto, molto più puntuale. Significa ancora affrontare il tema del bicameralismo perfetto e, sicuramente, la riforma costituzionale e la riduzione del numero dei parlamentari. Siamo pronti a partire da questo, ma anche da ciò che è stato prodotto nella scorsa legislatura da molti senatori e dai Gruppi parlamentari in questo ramo del Parlamento. Ma certo, se si vive il Parlamento come un impaccio invece di applicarsi alla fatica e alla responsabilità a cui è tenuto chi governa, si va in un'altra direzione. E allora - mi spiace dirlo - invece di un Presidente del Consiglio Capo dell'Esecutivo e delle Assemblee parlamentari ci ritroviamo cuochi, capponi e tacchini. Ma questa è un'altra brutta pagina che non avremmo voluto vedere perché offende la dignità dei singoli e quella delle istituzioni che essi rappresentano, tutti, e i loro poteri democratici. Vorremmo quindi che questi comportamenti, questi atteggiamenti, così come anche questi provvedimenti, non venissero più prodotti. Vorremmo che si affrontassero per materie organiche le riforme serie di cui il Paese ha bisogno e su questo

l'atto che stiamo discutendo è particolarmente importante e incide in modo sensibile sull'organizzazione dello Stato. Lo vedo in senso positivo e non rimembro il passato che non c'è stato. L'*iter* legislativo testimonia la laboriosa attività del Parlamento a sostegno di un'azione governativa volta a predisporre norme chiare per rendere più efficiente la macchina dello dello Stato, la macchina pubblica, mentre la spinta allo sviluppo tecnologico insita in tanti articoli del provvedimento è la rappresentazione plastica del ritardo che il nostro Paese ha nei confronti della modernità. Si dà oggi una spallata ad un certo modo di intendere il ruolo della burocrazia, che ha caratterizzato per lungo tempo il proprio rapporto con i cittadini presentandosi con volti - perché no? arroganti e molte volte inefficienti. Ce ne sono stati anche tanti capaci, ma la maggior parte però non lo è stata. avanguardia di sistemi di controllo politico sulle imprese e le libere iniziative, ora dispensatrice di favori di dubbia legittimità si trattava solo di far riconoscere diritti. Quanti favori ho sentito asserire di fare quando si doveva solo far rispettare il diritto delle persone! L'ho sentito con le mie orecchie e vissuto con la mia persona politica.

sindacalese?), tutelato, per così dire, dalla legislazione più ampia, contraddittoria e farraginosa del mondo, non ha

ad adeguare la legislazione e le strutture burocratiche di vasti settori statali alla sfida globale, che non è solo tecnologica, ma anche tra uffici pubblici snelli ed efficienti, tra chi è prigioniero di retaggi ideologici

certe inefficienze contenuto nell'articolo 22, con il quale, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare sul mercato i servizi

La legge in esame riguarda numerosi altri ambiti: dalla riforma di enti strumentali di vari Ministeri, a norme per favorire il turismo,

dei testi normativi e della pletora di leggi che affligge il Paese e che, come dicevo prima, è la vera grande protettrice di tutte le inefficienze.

che richiama interventi a favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, favorendo forme di flessibilità che possono essere particolarmente utili, specie alle donne, ma - lo ripeto - anche alle famiglie. Certo, la complessità delle problematiche affrontate richiederà una legge organica, in grado di riordinare e portare a sistema quanto già disposto in diversi provvedimenti, ma anche di risolvere in modo più globale e innovativo le questioni. strada della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro consentirebbe di raggiungere molti obiettivi. Mi appello dunque al Governo, e so che in esso vi è sensibilità sufficiente per accogliere quanto sto chiedendo, perché venga al più presto proposta una regolamentazione nuova e globale in tale ambito. Concludo sottolineando che a questo punto dell'*iter* legislativo è urgente varare al più presto e definitivamente questo disegno di legge. Voglio ricordare che non è un atto a sé stante, ma si raccorda a numerose altre norme, poste in attuazione, della legge finanziaria dello scorso anno e del programma di Governo votato dagli italiani. Il mio voto sarà pertanto favorevole. Grazie per l'attenzione, per avermi ascoltato e per la pazienza che avete dimostrato.

Abbiamo già avuto modo di sottolineare che la riforma, significativa, di buona parte del rito del lavoro

dell'azione collettiva. Non è quindi la prima volta che sottolineiamo, in Aula e in Commissione, questo modo un po' strano di procedere o perlomeno, dal nostro punto di vista, non condivisibile:

l'organizzazione della giustizia e, quindi, la possibilità di riforme vere ed efficaci che vanno in qualche misura ad incidere sui tempi dei processi e sulla

per quanto concerne il giudice deve essere indicato già nell'eccezione il giudice che si ritiene competente a giudicare la causa. Non vogliamo ricostruire tutto il provvedimento, perché oggi

rendere il provvedimento più efficace e pertinente alle finalità che si proponeva. Resta il grande interrogativo rispetto al metodo e alla procedura seguiti in questo anno

e forse, anche se sono state evocate nel corso dell'*iter* parlamentare, meritano qualche parola in più. Mi riferisco agli articoli 3, 4 e 5. 5. Sull'articolo 3 non posso che compiacermi per la conferma che la Camera dei deputati ha dato al testo del Senato condividendo, oltre il contenuto, anche una questione che non è di poco conto. La norma contenuta nell'articolo 3 prevede l'inserimento nella legge fondamentale in materia di produzione normativa da parte del Governo, la legge n. 400 del 1988, di una disposizione che impegna il Governo, nell'emanazione di norme di qualsiasi livello e rango (si citano

Proviene da una disposizione introdotta a suo tempo dalla Camera, che era per così dire indirizzata al vento, senza destinatario. Invece, con l'inserimento fatto dal Senato e condiviso dalla Camera è divenuta norma indirizzata specificamente al Governo, ma non è l'unica che

la preminente considerazione delle materie codificate e riordinate quando si effettuano interventi legislativi. Mi fa piacere che il Sottosegretario che assiste a questa discussione sia proprio quello per la giustizia perché uno dei produttori e dei destinatari del maggior numero di norme è proprio il suo Dicastero. Mi spiace sia momentaneamente assente il vice ministro Vegas, ma un altro Ministero interessato è proprio quello dell'economia. che essi stessi ed i loro uffici facciano mente locale a queste disposizioni che, mi auguro, tra oggi e domani diventeranno legge dello Stato. La seconda norma è quella riferita all'articolo 4 che interviene sul cosiddetto taglia-leggi, che è in dirittura di arrivo. Il 16 dicembre

che a tutto il 31 dicembre 1969 meritano di restare in vigore. Tutte le altre norme datate fino a quel momento e non citate s'intenderanno abrogate. Questo articolo Questo articolo organizza meglio l'effetto, così drastico, del taglia-leggi prevedendo, contrariamente al testo originario: che il 16 dicembre 2009 una verifica con i decreti legislativi ricognitivi; che successivamente, ove non vengano modificati, vi sia l'effetto abrogativo

una scadenza dei termini più ragionata, più meditata, più razionale che aiuterà senz'altro il percorso di questo modello di riordino del sistema legislativo molto drastico, drastico, ma per questo anche molto rigido, che viene in un certo qual modo ammorbidito. La Camera poi ha tradotto nell'articolo 4 una disposizione che recupera il decreto-legge n. 200 del 2008

Grazie conteneva una serie di norme di ratifica di trattati internazionali - il mondo del diritto internazionale è un po' a sé stante e questo fatto ha messo in agitazione non solo il mondo

la prima prevede che il Governo, con propri Regolamenti, quindi con attività tipicamente governativa, possa procedere alle abrogazioni e al riordino di regolamenti previgenti. Dagli accertamenti fatti in questi anni per il cosiddetto taglia-leggi si è verificato che il monte maggiore di norme è contenuto nei regolamenti governativi e ministeriali.

a riordinare, abrogare e riorganizzare tutto il sistema dei regolamenti, anche prescindendo da interventi legislativi. Il comma 2 di questo stesso articolo prevede, a regime, la possibilità per il Governo di produrre testi unici compilativi, cioè non innovativi delle leggi ma che mettano in ordine la legislazione esistente e quindi consentano agli operatori del diritto, alle famiglie, ai cittadini, ai professionisti, ai magistrati ed alla stessa pubblica amministrazione, di disporre di una fonte, quantomeno autorevole e qualificata, sulla quale poter far affidamento nell'applicazione delle leggi. A mio modesto avviso, una volta entrato in vigore questo collegato

riforma importante come quella del codice di procedura civile sia stata inserita in un collegato alla manovra finanziaria.

nonché in materia di processo civile». Si è cioè trattata questa riforma del codice di procedura civile come se fosse funzionale allo sviluppo economico del Paese. Paese. È stato anche detto che la riforma civile veniva fatta per favorire gli investimenti stranieri in Italia, quanto gli stranieri non vengono ad investire in Italia per la lunghezza del nostro processo civile. Guardate che le multinazionali e le imprese straniere che vengono ad investire in Italia hanno già provveduto per conto loro a porre rimedio ad una situazione

Qualsiasi avvocato che è in questa Aula sa perfettamente come ormai sono fioriti in tutto il territorio italiano studi associati di carattere internazionale in cui si richiede ai giovani che ne vogliano far parte di sapere perfettamente l'inglese e naturalmente anche di aver fatto *stage* all'estero, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, perché le clausole compromissorie riguardano proprio l'attribuzione della competenza a decidere di quelle controversie

un materia così importante come quella della riforma del codice di procedura civile alla Commissione giustizia? Eppure nella Commissione giustizia, anche da parte

le vere cause dei ritardi nella definizione dei nostri processi civili. È regola fondamentale che ogni volta che si deve affrontare e risolvere un problema bisogna conoscerlo a fondo. Per quale Per quale ragione le imprese straniere che vengono ad investire in Italia si vogliono sottrarre e si sottraggono con la clausola compromissoria alla giustizia italiana? Per il semplice fatto che i processi civili in Italia hanno una durata assolutamente inaccettabile.

relazioni o le relazioni inaugurali del presidente della Cassazione o dei vari presidenti della corte d'appello. Basta leggere l'ultimo rapporto *Doing Business* della Banca mondiale,

Gli avvocati sanno, come lo sa il sottosegretario Alberti Casellati qui presente, qual è la causa di questi grossi ritardi:

Paese ha un carico di cause del 40 per cento superiore a quello degli altri Stati. Non solo: è stato più volte scritto che il nostro Paese ha un carico di cause civili pari (pari!) a quello della Francia, della Spagna e di quasi tutta l'Inghilterra messe assieme. assieme. Questa è una delle cause principali. La seconda causa viene individuata nella pessima distribuzione dei magistrati sul territorio.

che non devono essere trattate contemporaneamente più cause poiché il giudice, che non è in condizione di conoscerle tutte, stenta ad impadronirsene e ad impedire i vari espedienti dilatori degli degli avvocati. Badate bene, anche gli avvocati sono in numero veramente spropositato rispetto ai giudici; i giudici sono meno di 10.000, gli avvocati sono 230.000. sono 230.000. Quindi, anche questo ha la sua rilevanza sulla possibilità di definire le cause. Un'altra causa che è stata individuata da altro gruppo di lavoro sempre in sede internazionale e universitaria è stata la rotazione dei giudici. Sappiamo benissimo che in alcune sedi, quelle disagiate cui accennava il collega Galperti, c'è una rotazione ogni due anni:vi

Inoltre, un presidente di tribunale intelligente, che si va a guardare - a differenza di noi in Parlamento - le risultanze delle indagini che sono state fatte, ha scoperto che se le cause si trattano a piccoli gruppi, quindi conoscendole, si fa molto

ossia l'ufficio del processo. Il senatore Maritati era Sottosegretario nella precedente legislatura e anche il Sottosegretario qui presente sa benissimo che nella scorsa legislatura si lavorò proprio a questo al Ministero,

dello stesso. Nella passata legislatura, il Governo di centrosinistra pensava che fosse indispensabile porre il magistrato in queste condizioni e quindi aveva pensato all'ufficio del processo, cioè un ufficio che potesse collaborare con il giudice perché arrivasse alla prima udienza in condizioni di conoscere perfettamente il processo e di governarlo: questo è l'importante per la definizione dei processi. Ma di tutto questo non abbiamo parlato.

che era una delle norme speciali. Noi l'avevamo detto: attenzione, se è vero che il carico di lavoro del magistrato è la causa principale della lentezza del sistema in modo che al magistrato arrivino pochi processi che possa decidere con grande velocità.

consente al giudice di convocare le parti solo per l'interrogatorio formale e, solo su sollecitazione, per la conciliazione. Perché non abbiamo modificato la norma

cioè gli uffici di transazione creati dagli avvocati che dovrebbero portare ad una definizione. Ciò peraltro a Monza sta funzionando perché gli avvocati si sono messi d'accordo avendo anche loro compreso che l'importante è fare arrivare al giudice il minore

per il giusto processo la prova dovesse essere raccolta davanti ad un giudice terzo e in contraddittorio.

conforme alla decisione: ciò urta infatti contro un principio fondamentale, che è quello dell'interesse ad impugnare una sentenza. Che interesse ho ad impugnare una sentenza che mi dà ragione e che è conforme alla giurisprudenza?

La giurisprudenza è difforme se la motivazione è diversa? Deve essere conforme alla conclusione; non ci siamo proprio. Così come non ci siamo con l'altra dichiarazione sulla violazione dei princìpi del giusto processo. Mi domando come si faccia ad

avevamo già espresso il nostro giudizio ampiamente negativo quando questo provvedimento è stato esaminato in prima lettura dal Senato. Giudizio negativo perché ritenevamo che la riforma della procedura civile - mi riferisco a questa parte del provvedimento fosse materia molto impegnativa, tale da richiedere un intervento di sistema e di struttura,

Ecco perché nella scorsa legislatura il Governo si era mosso nella direzione di provvedimenti armonici caratterizzati

dai provvedimenti più organici. Abbiamo preso qua e là alcune di queste norme prospettandole come riforma della procedura civile (la stessa cosa sta avvenendo per la procedura penale), affermando che si che si tratta della risposta che il nostro Stato dà alla crisi - che esiste - del settore della giustizia e che, com'è stato ricordato, è determinata dall'alto numero del contenzioso: ogni 100.000 abitanti, ogni anno entrano nel sistema giustizia, solo nel settore civile, 6.500 processi. Lo stesso numero di processi che entrano nel sistema giudiziario di Spagna, Inghilterra e Germania messe insieme. insieme. Questo dimostra che qualcosa del nostro sistema non funziona, per cui era necessario intervenire. Dopo aver fatto la solita ricognizione sulla giustizia che non funziona, sul ritardo della giustizia, bisogna interrogarsi sui relativi

la tipica legislatura in cui i grandi progetti di riforma potevano avviarsi con dibattito, discussione e confronto e portarsi al risultato. Ciò, però, non è avvenuto: non è avvenuto: ce ne dispiace perché è un'occasione persa. Per entrare nello specifico del provvedimento oggi al nostro esame in terza lettura, devo purtroppo sottolineare che proprio le conseguenze di questa visione non armonica

con un tratto di norme. Il nostro sistema da sempre - come tutti i sistemi di tradizione di diritto romano era impostato sul fatto che il precedente giurisprudenziale non costituisse vincolo per il magistrato e per il giudizio; potesse costituire un'indicazione, ma - ripeto a differenza dei sistemi di *common low* in cui il precedente giurisprudenziale viene equiparato alla norma.

che ci accingiamo ad approvare, invece, abbiamo inserito nel nostro sistema la promozione del precedente giurisprudenziale a livello di norma.

la cristallizzazione del diritto e della giurisprudenza. In tal modo, quindi, creiamo una supercassazione: creiamo una sezione che potrà stabilire se e quando è maturata l'ora x nel quadrante della storia giudiziaria per cui un precedente giurisprudenziale possa essere rivisto.

Il nostro sistema già prevede il regime delle inammissibilità del ricorso, che è interno al sistema di valutazione delle sezioni, le quali possono decidere se procedere in udienza pubblica o in camera di consiglio quando debba valutarsi sull'inammissibilità.

non offrono elementi per confermare o mutare la decisione. Vediamo cosa accade in questi casi: arriva il ricorso

per dichiarare l'inammissibilità. Quindi, l'apposita sezione creata non decide sull'inammissibilità, ma deve verificare se sussistono i presupposti. Questo

di cui all'articolo 376, cioè l'apposita sezione che dovrebbe giudicare sull'inammissibilità, se ritiene se ritiene che sussistono i casi di inammissibilità deve compilare una relazione per chiedere un giudizio in camera di consiglio. A quel punto il presidente della Corte, ricevuta questa relazione, fissa l'udienza in camera di consiglio per decidere sull'inammissibilità. In sostanza, abbiamo creato una sezione filtro che non decide, ma deve esclusivamente valutare in prima battuta; poi viene fissata l'udienza. l'udienza. Si è detto che questo sarebbe un metodo deflattivo delle pendenze dei ricorsi in Cassazione: è esattamente il contrario. Infatti, per un ricorso che attualmente potrebbe essere dichiarato inammissibile dalla sezione a cui viene assegnato, oggi invece ci vogliono due giudizi: un giudizio prognostico dell'apposita sezione e uno della sezione cui viene affidata la decisione dell'inammissibilità. Quindi - ripeto - un duplice giudizio sulla stessa questione.

sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni. Ma

che a comporre la sezione di cui all'articolo 376, ossia sezioni unite e singole sezioni, sono chiamati magistrati appartenenti a tutte le sezioni. Ma che significa? Che volete dire e cosa vogliono dire i colleghi della Camera dei deputati con questa norma? Forse che le sezioni semplici vanno costituite con componenti di tutte le altre sezioni?

il funzionamento della Corte di cassazione. Dobbiamo assumerci la responsabilità di ciò che intendiamo fare, al di là delle ragioni politiche secondo cui un provvedimento deve arrivare in porto assolutamente perché ciò è imposto La politica impone serietà nei comportamenti, nelle decisioni, nell'assunzione del proprio ruolo e nell'organizzazione di tale ruolo in funzione politica ma anche tecnica. Siamo chiamati a produrre, in funzione dei cittadini, leggi che siano leggibili, comprensibili e che non siano fonte di distorsioni radicali del nostro ordinamento, che abbiano un obiettivo contrario alla deflazione o che contengano assurdità tali da rendere incomprensibile e difficile

al di fuori di ogni razionalità normativa, un autentico bisticcio di volontà fra ciò che si assume di fare e ciò che si offre ai cittadini. Ritengo che il Senato possa,

credo che chi è intervenuto prima di me abbia già ampiamente sviluppato il tema di una quasi totale discrepanza tra i titoli con i quali partono questi convogli legislativi, rappresentati dai collegati alla legge finanziaria, e i contenuti reali con i quali arrivano a destinazione.

cioè destinazioni alle quali forse il macchinista o colui che muove gli scambi magari non ha voluto intenzionalmente condurre il convoglio,

di legge che il Senato esamina questa mattina, oltre a contenere norme sullo sviluppo economico, sulla semplificazione, sulla competitività e sul processo civile, aggiunge norme sul processo amministrativo e sul rapporto tra le giurisdizioni che avrebbero sicuramente

Ciò dovrebbe far riflettere sulla modernità e sulla capacità dei collegati di rispondere in termine di rapidità, ma anche di appropriatezza del lavoro legislativo al fine per cui furono

qualche apprendista stregone della tecnica legislativa ha introdotto una norma, che personalmente non riuscivo a capire, che riguarda la trasmissione e la comunicazione di documenti tra le pubbliche amministrazioni e, in particolare, alle alle amministrazioni di enti locali sotto i 5.000 abitanti. Una norma cioè che starebbe bene in una disciplina generale sul procedimento amministrativo, ovvero sulla trasmissione in favore di questi piccoli Comuni di flussi di informazioni in possesso di altre amministrazioni; ma cosa c'entra con la nuova disciplina delle farmacie? Vorrei citare come fatto oggettivamente pericoloso per il nostro sistema imprenditoriale e industriale, ma anche per la qualità della normazione, la continua autorizzazione di deleghe in materia ambientale. Sono quattro o cinque anni che queste norme si scrivono, si sovrascrivono, si cancellano e si scrivono un'altra volta. Vorrei dire - mi spiace che non sia presente in Aula un rappresentante del Governo nella materia specifica, ma credo che il sottosegretario Vegas riferirà riferirà - a chi amministra la cosa pubblica in materia ambientale, di non essere preda, di non mettersi a disposizione dell'ultima delle *lobby* che viene a chiedere la riscrittura della disciplina generale su questioni che attengono l'ambiente. Sono temi troppo delicati per essere lasciati al continuo moto di una risacca di *lobby* che si abbattono sugli uffici del Ministero dell'ambiente.

le leggi di questo Parlamento attraverso il sistematico attingere ai fondi per il Mezzogiorno, ai fondi per le aree sottoutilizzate e ai fondi CIPE, che abbiamo riprogrammato con atti legislativi. Ebbene, c'è una norma all'articolo 14 che impone a questi cattivi enti locali e a queste cattive amministrazioni regionali la cosiddetta tracciabilità finanziaria. Vuol dire che esse dovranno dichiarare, quando spendono dei soldi che derivano da queste fonti finanziarie, che sono derivati da lì, che li hanno presi in un determinato mese e li hanno utilizzati in un appalto, magari dopo sei mesi e non quattro, come dicono le norme stesse. insomma, far fare delle brutte figure alle amministrazioni lente; un sistema «brunettiano» per incitare la spesa corretta dei fondi che lo Stato mette a disposizione delle autonomie locali. Ma, allora, dovremmo dire a molti concittadini del Nord Italia: caro concittadino, tu oggi viaggi su questo treno perché questi soldi sono stati sottratti al tuo concittadino della Campania, dell'Abruzzo, della Calabria e della Sardegna; tu non paghi l'ICI perché abbiamo preso i soldi dalle aree sottoutilizzate. Questa tracciabilità che lo Stato chiede alle amministrazioni locali dovrebbe imporla, prima di tutto,

invece un'altra società, la IN.SAR spa che si trova in Sardegna, che viene liquidata, ma i posti di lavoro non sono garantiti e i danari derivanti dalla liquidazione - che provengono da leggi a favore delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno - vengono incamerati

trasfonde in un unico soggetto enti che oggi si occupano dell'informatica nella pubblica amministrazione e della formazione (la Scuola superiore della pubblica amministrazione); ma l'esito di questo processo non è indicato dal legislatore, ma dal Governo, al quale viene lasciata totale libertà di procedere come meglio ritiene.

un'idea di Parlamento che poi si trasforma nelle parole di inutilità e addirittura di dannosità che abbiamo sentito dal Presidente del Consiglio nei giorni scorsi.

nel delegare all'Esecutivo parti troppo grandi ed importanti della sua funzione. Non esistono criteri direttivi su questa materia; quelli che vengono chiamati princìpi e criteri direttivi non sono altro che la ripetizione insistita dell'oggetto della delega, mentre invece si attribuisce troppo al Governo quando gli si affida il riordino delle competenze del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni. Si sta dicendo cioè che il Governo stabilirà

della giurisdizione, che sono chiamati semplicemente a fissare un punto di interpretazione della legge, che è in definitiva la volontà del legislatore. Come farà il Governo di fronte ad un conflitto di giurisprudenza tra le sezioni della Cassazione o del Consiglio di Stato, o tra Cassazione e Consiglio di Stato, come avviene oggi? Proporrà alle Commissioni parlamentari un testo A e un testo B? Attenderà che si evolva la giurisprudenza di queste Corti superiori? Credo che non stiamo facendo bene il nostro lavoro: stiamo rinunciando a farlo. Ho concluso, colleghi. Vi chiedo: ma tutto ciò è solo un errore? È solo frutto di quei macchinisti impazziti, di coloro che fanno gli scambi al convoglio, oppure dietro c'è e non ve ne accorgete una ideologia che poi porta alle affermazioni sulla inutilità del Parlamento? Non è che qualcuno vuole farvi sbagliare, non vi accorgete dell'errore, ne diventati complici e poi, quando ve ne accorgerete, sarà troppo tardi? Noi, di questa complicità, non vogliamo essere responsabili. finestra"). Desidero informare i colleghi che è presente in tribuna l'onorevole Elena Espinosa, Ministro dell'agricoltura e dell'ambiente del Regno di Spagna, che ha partecipato al convegno organizzato dal Senato per promuovere la dieta mediterranea ed inserirla quale bene culturale protetto dall'UNESCO, in conformità della mozione recentemente votata all'unanimità dall'Assemblea del Senato a sostegno dell'iniziativa promossa dall'Italia insieme a Spagna, Grecia e Marocco. Al Ministro diamo il nostro benvenuto.

Su sollecitazione della Commissione europea è stata avviata la procedura di liberalizzazione del cabotaggio marittimo e di privatizzazione delle società esercenti i collegamenti marittimi per le isole per le isole maggiori e minori. Ci risulta che la società Tirrenia sarebbe aggravata, al momento, di 900 milioni di euro di debito e continuerebbe a subire una perdita annuale di 200 milioni di euro. Ciò nonostante, in base ai dati forniti dalla Corte dei conti, sembrerebbe che i compensi corrisposti all'amministratore delegato Franco Pecorini, alla guida della compagnia dal 1984, e agli altri amministratori

che una compagnia italiana non debba andare in mano ai soliti noti, e mi riferisco ad alcuni soggetti che già si sono fatti avanti, (privati che tanto privati non sono per la compagnia marittima, ma solo per le proprie

altresì contrari a queste categorie e organizzazioni sindacali, quali la CGIL, la CISL e la UIL, che invece di aiutare i marittimi li stanno penalizzando. Fortunatamente, insieme anche all'Italia dei Valori

i loro quotidiani soprusi che diventano ancora più odiosi se praticati a danno delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto. Non solo, come ho segnalato, la revoca dei fidi, o quella delle carte di credito da parte di una banca estera, la richiesta di tassi elevatissimi da parte di alcune banche operanti nell'Aquilano. Da un'indagine condotta da responsabili locali dell'emittente televisiva regionale abruzzese a TV7 è emerso che è emerso che il tasso d'interesse praticato da due grandi banche ai cittadini aquilani che hanno chiesto piccoli prestiti fiduciari finalizzati alla ristrutturazione dell'abitazione danneggiata dal terremoto varia dall'8,50 all'8,90

Le richieste ai cittadini aquilani e l'offerta dei due istituti di credito sono documentati dai filmati realizzati con una telecamera nascosta, di cui la prefettura del capoluogo ha chiesto di avere la registrazione. L'inchiesta è stata mandata in onda dalla trasmissione "Sotto le colonne", con riferimento ai portici dell'Aquila che storicamente rappresentano il salotto della città dove solitamente si discute di politica, cultura, sport ed attualità in genere.

questi comportamenti inaccettabili e vessatori del sistema bancario non devono essere più consentiti. E mi auguro che il Governo faccia una vigilanza preventiva visto che la Banca d'Italia

Grazie